2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche´

Grazie,

L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonche´ ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche´ altre disposizioni in materia di coesione sociale

un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno;

ad un’iniziativa abbastanza ambiziosa e costosa, cosı com’eformulato dal senatore Cioffi. La direttiva n. 27 del 2012, che dovremmo recepire nei prossimi due anni, contiene gli stessi temi, ovvero le stesse problematiche e gli

Prego,

Prego,

a valutare l’opportunitadi

sia nelle ganasce del Patto di stabilita. Chiediamo infatti che le proprieta pubbliche siano escluse dall’assoggettamento al Patto di stabilita. Non sembrava un

Le ditte che producono accumulatori sono per lo piu italiane ad altissima tecnologia. Oggi non si fanno questi investimenti perche´ hanno altissimi costi d’installazione. apparecchiature tra le previsioni delle detrazioni, potrebbe essere un nuovo sbocco per il nostro sistema industriale e per dare maggiore efficienza energetica alle abitazioni di nuova realizzazione. Pertanto, chiediamo la

sono eccessivi e addirittura non utili. Temiamo di aumentare complessivamente il costo del sistema.

ai Comuni. Intervenire sull’illuminazione pubblica non significa solo risparmiare energia, ma anche migliorare la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento luminoso e mettere a norma gli impianti fatiscenti.

Prego,

La bozza del decreto-legge prevedeva il termine di quattro mesi, mentre la Commissione ha proposto a maggioranza ed ottenuto la proroga a sei mesi. Ricadiamo, comunque, nel corrente anno di esercizio esercizio ed i Comuni e le Province sicuramente non hanno i soldi a disposizione, ne´ il tempo per occuparsi di questa cosa. Giacche´ i Comuni e le Province non hanno i soldi per provvedere alla manutenzione

l’emendamento 6.205, come altri presentati da altri Gruppi, ha l’obiettivo di estendere le agevolazioni non solo agli impianti termici, ma anche agli impianti tecnici della casa.

Come enoto nel momento in cui il privato o la societa intendono porre in vendita o mettere in locazione lo stabile o l’immobile sono obbligati ad indicare l’indice di prestazione energetica.

tende, da una parte, a mantenere l’obbligo in capo al mediatore di informare la parte della necessita dell’indicazione dell’indice di prestazione energetica nell’annuncio. Laddove peroquesto non dovesse accadere in maniera puntuale, nella seconda parte dell’emendamento si indica la possibilita per il mediatore di chiedere alla parte – persona fisica o societa– di sollevarlo dalla responsabilita relativa all’indicazione dell’indice di prestazione energetica, trasferendo, di conseguenza (come prevede la legge), la sanzione in capo al proprietario dell’immobile.

Grazie,

Signor Presidente, chiedo, a nome del Gruppo della Lega Nord di poter sottoscrivere, se il collega Gibiino e` d’accordo, l’emendamento 6.203. DALLA senatore Dalla Zuanna.

questo tipo di proroga aveva trovato attenzione e anche accoglimento, o almeno in parte del Governo: cosıera stato autorevolmente assicurato. Allora, io mantengo le decine di migliaia di utenti e di associazioni che, giustamente, fanno il loro dovere, segnalando al Parlamento le difficolta che possano insorgere con provvedimenti immediatamente attuativi, 2013 vano situazioni che invece, con un po’ di buon senso, si spalmano nel tempo. Proprio per trasparenza e linearitaio mantengo l’emendamento, sperando che, nel corso ulteriore di questa vicenda parlamentare, e nel caso esso fosse bocciato, possa essere corretto un no che, evidentemente, non viene adeguatamente motivato rispetto a giuste esigenze che una categoria rappresenta nel momento in cui va ancora piu in crisi, ed e` peraltro un comparto fondamentale della nostra economia.

Passiamo quindi alla

Dovremmo fare una revisione di questi tasti!

senatore Di Biagio). il testuale recepimento degli articoli 6 e 7 della direttiva 2010/31/UE, attraverso l’inserimento corretto della cogenerazione quale sistema alternativo ad alta efficienza. Tale riferimento consente di declinare nella maniera piuidonea l’attuale recepimento delle disposizioni relative alle procedure di installazione e di utilizzo di unita di cogenerazione, a partire dalle unitadi microcogenerazione ad alto rendimento, gia rispondenti alle direttive comunitarie, alimentate a gas naturale. Tale tipologia di installazione e di impiego determina notevoli risparmi in termini di energia primaria

parte delle disposizioni indicate dalla direttiva comunitaria: cio potrebbe consentire di raggiungere i livelli di avanguardia di Germania e Gran Bretagna, promuovendo a costo zero un importante piano di efficienza energetica degli edifici che si pone strategicamente in linea con l’attuazione delle disposizioni previste dal piano casa, degli interventi di ristrutturazione urbanistica e del piano per le citta`.

Ritiro l’emendamento 12.4.

Robin Tax – tutti i soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego di fonti rinnovabili.

che alcune Regioni e Province autonome hanno gia emanato notificando i relativi atti alla Commissione europea. In questo senso enecessario un aggiornamento ad una clausola gia esistente nel testo del decreto legislativo in vigore.

confesso che ho qualche difficolta` a comprendere le ragioni della richiesta. Se mettessimo un riferimento alla mancanza di oneri aggiuntivi e la formula: «nell’ambito delle risorse disponibili», forse potremmo risolvere il problema e mantenere anche il primo comma

Avverto inoltre che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento 15.0.500, trasmesso dall’Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza parere non ostativo. DI BIAGIO

l’emendamento 15.200 intende sostituire completamente l’articolo 15 del provvedimento in esame, prefiggendosi di declinare in maniera opportuna la realizzazione di programmi di ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica, di risparmio e di efficienza energetica del patrimonio immobiliare nei settori civile, del terziario, industriale e agricolo, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, di mobilitasostenibile, oltre che di ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio. In particolare, si propone l’inserimento della proroga degli ecobonus nel decreto-legge di recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero quale occasione di rilancio della riqualificazione urbana e del territorio, nell’ottica di istituire un fattivo collegamento tra gli interventi di riqualificazione di unita immobiliari, piano casa e piano di governo del territorio improntati alla sostenibilitaambientale attraverso interventi orizzontali di ristrutturazione urbanistica. Inoltre, si interviene affinche´, a partire dal 2014, l’attuale regime di incentivazione in ambito edilizio ed energetico venga indirizzato alla realizzazione di una rete tra le diverse misure fiscali e gli strumenti finanziari, attivando un fondo rotativo ad hoc accessibile ai soggetti certificati che, nel ruolo di investitori, sollevino il cittadino cliente finale, ormai sempre piu in difficolta` economiche, dall’investimento.

15.5 estato trasformato in un ordine del giorno,

Questo non determina il superamento del parere contrario della 5ª Commissione, anche se lo presenta il Governo; anzi, dovrebbe presentare anche la relazione tecnica.

Quindi questo emendamento, se approvato quello successivo, poteva essere assorbito anche come ordine del giorno. Sull’ordine

del Governo vuole rispondere subito, cosı` da esaurire l’argomento?

l’aumento delle tipologie e irrilevante, essendo salvaguardato il tetto previsto. Quindi, anche con quella formulazione si puo` votare.

sia meglio preferire il concetto di valorizzazione dello stesso, e le ragioni sono evidenti: noi non tuteliamo i settori, valorizziamo la loro possibilitadi sviluppo. Inviterei a considerare questo approccio, che non e assistenziale

il parere diventa contrario, perche´ questo ordine del giorno etroppo limitativo ed indica una prospettiva molto

Il relatore

La parte iniziale, quella sul sostegno all’industria del mobile nelle modalita previste econdivisibile, ma se la parte dispositiva, su cui mi ero rimesso, rimane nel testo attuale il parere e contrario.

(M5S). Signor Presidente, rimaniamo sbigottiti davanti a termini utilizzati dal sottosegretario Vicari nei confronti del Gruppo Movimento 5 Stelle! (Applausi dal Gruppo M5S). Per cui chiedo che immediatamente il Sottosegretario si scusi per le parole proferite.

5 Stelle. PRESIDENTE. Senatore Santangelo, credo che l’immagine che abbiamo trasmesso all’esterno delle istituzioni e del Senato non abbia bisogno anche di questo ulteriore elemento.

Stanno terminando gli incentivi sul conto energia e questo sarebbe un modo per completare un’opera di bonifica assolutamente fondamentale per il nostro Paese. Per questo mi permetto di insistere per la votazione. PRESIDENTE. Invito il

il sottosegretario Baretta ha invece espresso parere contrario. Senza voler ledere il principio di uguaglianza e sottolineando il fatto che i beneficiari della detrazione per l’acquisto di arredi sono quelli che hanno in corso la ristrutturazione edilizia, noi, sia per incentivare il settore del mobile arredo, sia per andare incontro alle famiglie e alle coppie che si sposano onde evitare di ampliare a tutti la platea dei beneficiari, avevamo proposto che tra i beneficiari ci fossero le coppie sposate dal 1º gennaio 2013. Questo eil senso e dell’ordine del giorno. VICARI,

di dare un termine alle riformulazioni. Giane vediamo alcune decine per articolo; poi ci viene imputato magari qualche ritardo o anche qualche imperfezione. Cosı ci emolto difficile lavorare. Noi siamo assolutamente collaborativi, pero lei comprende che dobbiamo riesaminare un certo numero di emendamenti. relatore. Signor Presidente, credo che il presidente Azzollini abbia posto un problema oggettivo cui mi associo e mi permetto di proporre una sospensione – anche breve, di trenta minuti – perche´ abbiamo bisogno, sia sui testi accantonati che sugli ultimi articoli, di coordinarci in maniera da terminare in tempi rapidi.

Senatore Bocchino, le

Voglio soltanto far notare che nel caso dei piccoli paesi o delle periferie delle citta` le edicole che distribuiscono gli allegati alle pubblicazioni e ai periodici rappresentano molto spesso l’unico canale di diffusione, in mancanza di vere e proprie librerie. quindi oltremodo penalizzante che si aumenti l’IVA sui cosiddetti allegati, in quanto questi costituiscono per una parte della popolazione l’unico canale per venire a contatto con supporti digitali, tipo i CD,

delicato. Infatti, e preoccupazione condivisa che l’aumento dell’IVA, in particolare sui prodotti editoriali legati alla scuola, al mondo dello studio, all’universita,

un ordine del giorno che invita il Governo a valutare la distinzione tra le due tipologie, noi lo accoglieremmo.

soprattutto per un Governo che ha esordito con l’impegno formale del Presidente del Consiglio a non procedere a tagli diretti e/o indiretti (e questo sarebbe il caso) al settore dell’istruzione e della cultura.

a convergere tutti sull’ordine del giorno G19.101 (testo 2): altrimenti siamo costretti a dare un parere negativo su un emendamento per poi accogliere un ordine del giorno che gli assomiglia.

andremo a cercarlo a palazzo Chigi.